il fatto che per molti colleghi, essenzialmente della maggioranza, del PD, la questione sia stata risolta come una semplice applicazione normativa, anzi, diciamolo pure, come un'operazione di necessità virtuosa per poter modificare il nostro ordinamento secondo i *desiderata* dell'Unione europea, che invece è sempre molto più attenta e avanti.

perché probabilmente non ha ancora realizzato il fatto di essere totalmente indifferente rispetto ai *desiderata* che stanno dietro a questo decreto-legge.

di aver dovuto adottare un decreto-legge per impedire speculazioni e per evitare che il mercato potesse creare anomalie: le abbiamo viste queste anomalie, Presidente, con le speculazioni fatte nei giorni successivi! Addirittura, in alcuni casi, come quello della Banca dell'Etruria, con crescite del 60 per

perché o non hanno capito cosa stanno facendo o non hanno capito la parte che stanno recitando. Sono molto arrabbiato per questo, perché i cittadini all'esterno ne sono tenuti all'oscuro e ancora una volta questa viene fatta passare come una riforma quando di riforma qui dentro non c'è nulla! Vengono al contrario soddisfatti interessi di parte, con un Presidente del Consiglio dei ministri che abusa degli organi costituzionali: il Senato non ha avuto tempo nemmeno di svolgere un lavoro serio in Commissione,

signora Presidente, non occorreva essere degli scienziati per andare a leggere, nei giorni passati, alcune dichiarazioni dell'amministratore di Unipol Gruppo Finanziario e UnipolSai, Carlo Cimbri, come riportate dalla stampa. Si legge, su «Milano Finanza» quest'ultimo ha espresso parole di grande apprezzamento per il provvedimento sulle banche popolari fortemente voluto da Renzi, sottolineando: "regole di *governance* uguali per tutti sicuramente costituiscono una correzione" e che "viene corretta un'anomalia che certamente innescherà processi di aggregazione. Sotto questo profilo, condivido la posizione del legislatore che condurrà ad un riassetto del nostro sistema bancario".

che è Unipol Banca, finalmente Unipol Gruppo Finanziario ne prenderà il controllo, potendo così, finalmente, completare quel percorso e dire «abbiamo una banca»! Questo è quello che sta succedendo e mi rivolgo ai colleghi del Nuovo Centrodestra: cosa state sostenendo? Questi si stanno appropriando delle banche popolari, addirittura con la sfacciataggine di chi con un provvedimento di legge vuol farlo passare come riforma virtuosa per il sistema creditizio,

far passare come riforma qualcosa che invece serve per stabilizzare alcuni equilibri e una fame di denaro dall'estero. Le riforme bancarie si facciano a partire dalla separazione bancaria! L'abbiamo proposto più volte e ancora in Commissione e proprio oggi il Governo si è messo di traverso. Si parta da questi aspetti per riformare seriamente e tutelare il risparmiatore dallo speculatore. Altrimenti saranno per l'ennesima volti fondi accaparrati alla speculazione, per poter consentire dei giochi di potere. Ci piacerebbe

Quanti di quelli che voi oggi, con il vostro voto, finanzierete! E poi non stupitevi se, nel momento in cui vi saranno delle indagini, salterà fuori che ci sarà stata ancora qualche concessione, come quelle autostradali, in cui gli amici degli amici se ne sono avvantaggiati. Pensiamo a quello che sta succedendo qui dentro (e lo dico a voi, colleghi del PD): non potete far passare questa come una riforma delle banche popolari, perché questo vuol dire solo soddisfare degli appetiti politici e dei giochi di potere che garantiscono

Voi oggi non potete più dirvi difensori del popolo, ma solamente di *lobby* che vi stanno dietro e che, tramite le proprie capacità di pressione, vi obbligano a votare queste schifezze fatte dal Governo. sono strabiliato dal vedere la superficialità con cui è stato affrontato il tema, soprattutto oggi, nel giorno di scadenza del decreto-legge. Si potevano esaminare gli emendamenti e si poteva approfondire il tema. Certo, senatrice Ricchiuti, è vero che ci sono state negli anni delle gestioni non ben fatte sulle banche popolari, eccome se ci sono Ma questa non può essere una scusa per fare questo tipo di scempio, perché c'è una modalità operativa e c'è una storia delle banche popolari che non possiamo cancellare. Questo è quello che ha reso differente questo tipo di credito rispetto alle SpA e a quello che hanno fatto negli anni.

sappiamo che il Governo ne farà carta straccia fra qualche minuto, perché chiaramente ha portato la situazione a tal punto da obbligare per se stessa la fiducia. No, questo non è serio: questo vuol dire mancare di rispetto nei confronti dei cittadini e, ancora una volta, impedire che la politica faccia il proprio corso in maniera positiva.

penso che la discussione su questo provvedimento debba prescindere, almeno parzialmente, dal merito. Le

se sia cioè utile al Paese superare quella dimensione giuridica e anche quella modalità operativa di questa parte del credito o se sia. Dico che bisogna superare un po', almeno parzialmente, il tema del merito e concentrarci poco poco di più sul tema del metodo.

in legge e quindi, dovendo il Governo e la sua maggioranza difendere la possibilità di conversione, toglie al Senato, ai senatori, a questa parte di popolo rappresentato, di intervenire sul merito, cioè sulle singole disposizioni in esso contenute. Vale il ragionamento sul metodo anche per quanto attiene alla natura di questo provvedimento sotto il profilo costituzionale, costituzionale, cioè alla coerenza di questo provvedimento rispetto alla norma costituzionale che regola i decreti-legge.

il Senato e il Parlamento siano chiamati a decidere della costituzionalità o meno di un decreto-legge se questo lo si fa sulla base di un ragionamento politico e dei numeri della maggioranza? Lo sappiamo tutti; lo sanno i i colleghi della maggioranza, come lo sanno i colleghi dell'opposizione che hanno sostenuto le pregiudiziali: questo decreto è sotto il profilo costituzionale chiaramente ricorrono, infatti, le condizioni di necessità e urgenza ed è palese che non ricorrano queste condizioni per i tempi di attuazione che in esso sono contenuti, per l'articolazione dei temi che tratta e per il modo con il quale è stato scritto e proposto all'esame del Parlamento. Vale contestualizzare questo intervento.

reca scandalo. Siamo in un'economia di mercato e l'economia di mercato prevede che i soggetti economici possano essere scalati, cambiare proprietà e diventare un'altra cosa rispetto a quella che erano addirittura cambiare le finalità stesse della loro missione. Il problema è un altro e va contestualizzato rispetto a tutti i provvedimenti che riguardano l'economia, ma anche la riforma sul piano istituzionale. C'è un'idea che io non condivido perché non penso porterà bene al mio Paese. C'è l'idea della concentrazione e della centralizzazione dei poteri. Questa idea, che si manifesta nei provvedimenti che riguardano l'economia e in quelli che riguardano l'organizzazione sociale e istituzionale del nostro Paese, non attiene alla sola dimensione nazionale. Non si tratta neppure di sostenere o difendere le possibilità e le prospettive di poteri economici e finanziari oppure politici e sociali che sono all'interno del nostro Paese. Qua si tratta di fare qualcosa di più. Si tratta di definire la natura della sovranità di questo Paese in questi argomenti, come negli altri, che trasformano l'Italia da un Paese fondatore dell'Unione europea a un Paese comprimario di qualche Paese europeo in fase espansiva. Si tratta, cioè, di sottostare a poteri economici internazionali che intervengono ormai esplicitamente e senza farne alcun mistero. Le intercettazioni dei capitali esteri sono una delle cose che vantiamo di più come dato positivo. Lo si fa nell'industria; non si capisce perché non lo si debba fare nel settore finanziario. Ma se tutti questi poteri economici controllano la nostra informazione, influiscono nella nostra politica e assoggettano le nostri condizioni sociali ai loro meccanismi di sviluppo, alle loro finalità di profitto, se tutto questo avviene, mi chiedo quale sia il destino della nostra comunità e del nostro popolo. se sia chiaro in mente quali sono e quali saranno le conseguenze dei singoli atti - tutti ben fatti rispetto a quell'obiettivo - posti in essere dal Governo e dalla maggioranza. È da anni che ci facciamo dire dagli economisti come deve funzionare un Paese, come deve funzionare l'Unione europea, come dobbiamo regolare i rapporti sociali. che subiamo le ricette che ci vengono somministrate da questa *élite* di grandi pensatori. E io sarei contento di vedere un risultato per cui, se un padre di famiglia perde un posto di lavoro, sono due a conquistarne uno a testa, così come ci raccontano. Così come sarei contentissimo di vedere il prodotto interno lordo decollare e sarei ancora più contento di vedere i risultati della nostra economia condizionare positivamente la vita dei cittadini della nostra comunità. Ma questo non avviene, purtroppo. Passeranno di mano le banche popolari. Può darsi che le nostre piccole e piccolissime microimprese non accedano a nessun tipo di

E può anche darsi che alla fine di tutto questo percorso la crescita che noi vorremmo agganciare non si agganci affatto. Può darsi che abbia torto io può darsi che abbiano ragione tutti quelli che ci hanno insegnato come dovevamo comportarci fino ad oggi, anche se i dati non confortano quelle tesi. Presidente, almeno ci si consenta di discutere nelle Commissioni di merito, di approfondire gli argomenti. Che non si passi attraverso il trucco della decretazione d'urgenza e del voto politico sulla costituzionalità dei provvedimenti. Che si dia cioè la possibilità a noi tutti di ragionare sulle conseguenze, perché quelle conseguenze non le paghiamo noi, ma le pagano i cittadini e l'Italia!

relativamente all'Atto Senato 1813, ho visto che il vostro Presidente del Consiglio è andato in giro a farsi molta pubblicità: molto fumo per nascondere quel poco di cattivo arrosto che c'è dentro.

Dichiarazione del vostro Presidente del Consiglio: «Ci sono troppi banchieri e poche banche che prestano soldi». E infatti andiamo ad uccidere il comparto che presta soldi: le banche popolari. Come dice il Centro studi della CGIA di Mestre,

Inoltre, le banche popolari nei momenti di crisi prestano soldi, mentre le banche SpA tendono a rientrare dei loro prestiti. Quindi, le banche popolari fanno esattamente quello che bisognerebbe fare quando c'è crisi,

mentre le banche SpA hanno ridotto gli sportelli e così ridotto l'occupazione. Quindi, voi andate a colpire un settore che crea occupazione, cercando di trasformarlo in un tipo di banca che distrugge occupazione. Complimenti: zero su tre.

sono la gran parte; le altre 60 sono irrilevanti. Come sempre, però, basta citare solo un numero e non l'altro per far sembrare una cosa invece di un'altra. Per quanto riguarda gli attivi del Banco Popolare,

detto. Le banche popolari, dove uno vale uno (sono riuscito a dirlo), cioè dove ogni azionista rappresenta un voto, a prescindere da quante azioni possiede,

Oppure basta limitare il numero di volte in cui si può essere eletti a far parte del consiglio di amministrazione. Tutto questo si può fare per via statutaria: non c'è bisogno di andare giù con la motosega quando si può fare una cosa molto più semplice. Ma voi non l'avete fatta. Perché? Perché le banche popolari hanno un'altra peculiarità: sono le banche che, rispetto al prezzo di quotazione azionaria (quelle quotate), hanno il più alto valore patrimoniale, cioè sono quelle più ricche, dove ogni azione è quella che vale di più. Allora, niente di meglio che darle in pasto a quelli le cui azioni valgono carta straccia, tipo il Monte dei Paschi di Siena,

Bene, voi cosa fate? Costringete addirittura queste banche, che sono protette, ad andarsi a quotare. Un colpo di genio: regaliamole a qualcuno. Bene, regalarle a qualcuno cosa vuol dire? Oltre ai già citati motivi patrimoniali ci andiamo a prendere la cassaforte in una banca popolare che, per sua natura, è sottoquotata rispetto alle altre), le possiamo anche regalare ai contendenti esteri. Ricordo che i contendenti esteri sono sempre alla ricerca di questo tipo di grossi affari. Cosa otterremmo? Una riduzione dei posti di lavoro. Infatti, tutte le volte che si sono che si sono create queste aggregazioni bancarie, si è licenziata della gente. Infatti, se tu hai uno sportello, ad esempio di Unicredit, e a 50 metri hai uno sportello di UBI Banca, che te ne fai di due sportelli così vicini? Lo chiudi. Si chiama razionalizzazione e non è neanche stupido. È però stupido pensare di farglielo fare. Infatti, se vogliamo salvaguardare il lavoro non possiamo fare questo genere di stupidaggini. un'altra cosa. Voi dite che le popolari non sono radicate sul territorio. Ciò è falso, perché, anche se sono presenti in un gran numero di Province, esse sono comunque sempre espressione di un azionariato locale e prestano alle persone del territorio. Anche questo è un dato di fatto. Almeno cercate di portare dei buoni argomenti e non delle menzogne a sostegno di quello che dite. Qual è la seconda sorpresa dentro l'uovo? Ci sono due sorprese cattive. La sorpresa è che voi create una società veicolo che serve per aiutare le aziende che sono in difficoltà patrimoniale. Avete aggiunto anche industriali e a vocazione internazionale. Per questo motivo, giustificate l'uso della SACE, che è il braccio destro della Cassa depositi e prestiti e si occupa dell'internazionalizzazione. Che cosa vi viene in mente? A ma un nome solo: ILVA. Quindi, questo sarebbe l'ottavo decreto salva ILVA. Avete creato la società veicolo per dare soldi all'ILVA. Chi può mettere i soldi qui dentro? I privati. Però i privati con garanzia dello Stato. Bello quando uno investe i soldi e lo Stato garantisce! E poi possono farlo anche gli investitori istituzionali. Chi sono questi misteri? Gli investitori istituzionali non sono privati, sono anche il pubblico. Infatti avete scritto «enti previdenziali». Ma sì, un bel colpo di mano anche sulle casse previdenziali. Grande idea. Oppure l'INPS e la succitata Cassa depositi e prestiti, con la scusa che quest'ultima dovrebbe cominciare a fare del credito. Ma questa è una cosa vera dentro una cosa falsa. Non è questo il credito. Quanti soldi andranno in questa cassaforte? 300‑400 milioni, ma anche 500. Allora, sono 500 i milioni che potrebbero avere l'intera garanzia dello Stato a favore dell'ILVA di Taranto. Almeno lo aveste scritto! Il resto, quello che avete inserito, è fumo. Avete parlato di portabilità dei conti correnti (tre pagine di specifica), oppure di *start up* innovative, che vanno bene, buttando qualche milionata. Oppure avete parlato di conti transfrontalieri. Questo servirebbe per attirare gli investimenti esteri? Questo non serve. Allora, una volta tanto, dovreste avere il coraggio di dire perché fate le cose. Le fate perché volete regalare le banche popolari? Le fate per aiutare il Monte dei Paschi di Siena? Basta dirlo: sì, non vogliamo far fallire il Monte dei Paschi e lo facciamo per quello. Ditelo. Oppure la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio: potreste chiedere al papà della signora Boschi *(Applausi

le banche di credito cooperativo sono un intermediario chiave nel sistema bancario mondiale: sono 3.700 le banche di credito cooperativo, che a voto capitario si esprimono e si autoregolano

che sviluppano la loro attività e formano i loro attivi e i loro patrimoni. Secondo uno studio della Bundesbank, che se ne intende di banche popolari, popolari, nel sistema europeo vi erano 1.200 istituti e 13.600 sportelli regolati da principi mutualistici e di interesse sociale, con un bilancio aggregato di circa 1.000 miliardi di euro, al servizio di 30 milioni di clienti. Ad esempio, in un Paese come il Canada, l'importante banca Desjardins ha un attivo di 223 milioni di dollari canadesi, 45.000 addetti e 5,6 milioni di soci. Questa banca viene definita da Bloomberg - non dalla Lega della cooperative - la principale e la più solida banca del sistema nordamericano, in un'epoca in cui in quei Paesi la crisi ha picchiato pesantissimamente e la seconda banca del mondo. Questa è la realtà di oggi e questi sono i grandi numeri di oggi. Per tornare invece alle radici, dobbiamo molto a uomini che forse non tutti ricordano, come Schulze-Delitzsch o Guglielmo Raiffeisen e con loro l'italiano Luzzatti, che furono i fondatori delle unioni cooperative del credito bancario, tracciando i solchi nella terra in cui si svilupperà quell'economia sociale di mercato, frutto del fecondo intreccio di pensiero politico liberale,

animato da uomini e donne come Terracini, Togliatti, Malvestiti, Cortese, Fanfani, Taviani, dall'eccellente relatore dell'articolo 45 sulla cooperazione, il socialista Canevari, erede di Bruno Buozzi, da Lina Merlin da altre donne (quelle poche donne, ma dal grande peso sociale e politico, che animarono il dibattito sulle grandi questioni economiche e in particolare sulla cooperazione). È un ricchissimo dibattito quello che si sviluppa tra il 1947 e il 1948, che traccia il solco

assistite quasi esclusivamente dal credito mutualistico locale. Senza quel credito non avremmo avuto quelle imprese e non avremmo l'ossatura e l'architettura del sistema economico italiano. Il testo che ci consegnano i Costituenti, quindi, esalta nella libertà di impresa la cooperazione quale metodo democratico per fare impresa alternativa a quel sistema capitalistico puro. Cosa era quello della Costituente: un processo al capitalismo? No, era di più: è il processo ad una libertà, che della libertà non aveva che un volto menzognero, perché aveva solo garantito la libera sopraffazione gabellata per libera concorrenza. Così dichiarava Malvestiti in quel dibattito. Ma ancor più moderno, e più attinente alla realtà che viviamo noi oggi, è il contributo a quel dibattito del liberale Cortese, quando ricorda che se c'è una rivoluzione liberale da compiere - lo dico soprattutto rivolgendomi ai banchi del Gruppo al quale appartengo nel campo dell'economia, ed è diretta a ristabilire l'economia di mercato contro le degenerazioni capitalistiche, contro i cartelli, contro i *trust*, contro i *pool*, contro i monopoli di ogni tipo. Oggi, a quelle definizioni, noi possiamo solo aggiungere quella di intermediari finanziari, che ancora non era nota, che sovente, agendo da sedi in paradisi fiscali, muovono acquisizioni ostili per assorbire valore economico costituito nel tempo e bruciarlo nel falò della finanza della *deregulation* anglosassone. Con questo decreto volete compiere esattamente questo: rendere contendibile a quel modello di finanza l'intreccio fertile tra impresa cooperativa-banca e impresa diffusa sul territorio, che ha sostenuto con pazienza proprio quello sviluppo. Complici anche di vigilanze burocratiche asimmetriche, occhiute con alcuni e molto distratte su altri, come è già stato detto in quest'Aula, oggi votate contro la Costituzione italiana, che non consente che si imponga un limite, sia esso riferito all'ambito delle attività nelle quali la cooperazione può operare, sia che venga rapportato alla dimensione che la cooperazione può assumere. Questo all'interno di quel dibattito, un po' stupido, tra gli otto miliardi e i 30 miliardi; quei 30 miliardi stabiliti dall'Unione europea, che noi invece fingiamo di non vedere perché è più comodo al decreto di questo Governo concentrare la propria attenzione su quel limite per rendere ancor più possibile il processo di esproprio. Tutto questo ce lo ha ricordato Cesare Mirabelli Mirabelli - semplicemente un Presidente emerito della Corte costituzionale - in un suo commento ai lavori della Costituente, che spero aiuti voi (come ha aiutato me) a valutare con grande preoccupazione gli effetti di una legge che distruggerà economia, per arricchire il tragico elenco delle speculazioni finanziarie, ai danni di popoli non tutelati dai loro Governi e di sistemi economici sbranati dalla finanza più speculativa, come se la crisi del 1929 e quella del 2008 non ci avesse insegnato nulla. Ma non è stato così per tutti. Infatti, quando le BCE pubblicò lo scorso anno l'elenco delle 120 banche europee che sarebbero finite sotto la vigilanza unica, emerse rumorosamente, nella totale distrazione italiana, l'assenza di mezza Germania bancaria: 1.700 banche su 3.532 tedesche non superano la soglia sistemica, grazie a quel regolamento che citavo prima. Tra queste, tutte le casse di risparmio, tutte le cooperative, siano esse *Volksbank* o *Raiffeisenbank*, cioè quelle banche che sul territorio operano, crescono ed erogano credito grazie al principio del voto capitario nell'organizzazione della mutualità, prevalente e non prevalente. Questa è l'ossatura, il terzo pilastro del sistema bancario tedesco, che è il più forte d'Europa.

in Italia (nemmeno in Francia accadrebbe mai), si decreta l'esproprio della libera proprietà organizzata nella cooperazione verso la speculazione internazionale; tradotto, significa far risucchiare il risparmio, il ricco risparmio degli italiani (terzo risparmio al mondo), ancora detenuto nelle banche popolari, da quegli strumenti che chiamiamo alternativamente *hedge funds* o intermediari finanziari, che sembrano neutri ma non lo sono affatto.

Il presidente Grasso porta due grandi responsabilità in questo decreto. La prima è l'aver firmato un decreto‑legge totalmente incostituzionale: ma io sono serena, la Corte costituzionale si incaricherà di svergognare Governo e Parlamento, dichiarandolo incostituzionale.

che nei pochi giorni disponibili firmasse questo decreto, giacché né Napolitano, né tantomeno Mattarella avrebbero mai potuto firmare un decreto-legge che renderà più poveri gli italiani.

di quella Costituzione italiana della quale, invece, questo Governo e questa maggioranza faranno scempio.

su questo provvedimento si è svolto un dibattito molto acceso e molto intenso, in particolare con riferimento all'articolo 1, relativo alla riforma della banche popolari; una discussione interessante, certamente, anche se caratterizzata, in alcuni casi, da molte affermazioni - lo abbiamo sentito anche questo pomeriggio - poco rispondenti ai dati di fatto e, in qualche modo, molto lontane dalla realtà dei mercati odierni. allora, riprendere alcuni di questi temi, ma con una premessa, di cui ho sentito parlare poco o quasi per niente. quello che sta succedendo a livello internazionale e a livello europeo vogliamo parlare o facciamo finta di essere un Paese isolato da tutto il resto del mondo? A livello internazionale ed europeo sta avvenendo una vera e propria rivoluzione sul fronte dell'organizzazione dei sistemi di intermediazione finanziaria. È una rivoluzione - senatrice Bonfrisco - proprio per rispondere a quella crisi della finanza creativa e della leva finanziaria senza limiti che ha portato alla crisi del 2008-2009. I regolatori di tutto il mondo, in particolare quelli dei Paesi avanzati, sono impegnati sulla solidità delle banche ed in particolare sulla robustezza del loro capitale. Naturalmente, si può essere d'accordo o no su questi provvedimenti, ma non possiamo disconoscere che l'asticella si sta spostando sempre più in alto, ovvero che le singole banche vengono giudicate in grado di fronteggiare l'emergenza, e quindi le crisi, con il criterio chiave della capacità, in qualche maniera, di irrobustire e rafforzare il loro capitale, proprio per evitare quello che è successo in questi ultimi anni. anni. Su questo sfondo, vorrei parlare del provvedimento e rispondere ad alcune delle affermazioni che ho sentito fare questo pomeriggio.

Credo che molti interventi, anche quelli che mi hanno preceduto, abbiano chiarito che questo provvedimento del Governo non mette assolutamente in discussione il valore del modello delle banche popolari e cooperative, ma stabilisce qualcosa di importante. Questo modello non si addice a banche la cui dimensione supera un certo limite o che siano quotate in Borsa.

le vere banche cooperative popolari che mantengono questa natura possono conservare le loro caratteristiche e quindi continueranno ad operare. Le banche di cui parliamo e di cui si stabilisce la necessità di modificare lo statuto sono banche con peculiarità che ne fanno a tutti gli effetti delle vere e proprie grandi banche commerciali. Voglio ricordare queste peculiarità: la distribuzione di dividendi e l'utilizzo di utili, che ha una finalità del tutto analoga a quella delle banche e delle società per azioni; la possibilità di quotarsi in Borsa, che in qualche modo (come sappiamo) riguarda gran parte delle banche interessate alla riforma; la loro estensione su tutti i territori: non ha senso parlare ancora di relazioni con il singolo territorio, quando sappiamo, ed è stato ricordato

del modello cooperativo storico, quello radicato nelle tradizioni di origine socialista o cattolico-sociale del XIX secolo, a queste banche popolari resta soltanto un elemento: il voto capitario, con tutto ciò che sappiamo indebolisce la loro *governance*. Quello che il provvedimento ci dice, allora, è che queste banche popolari più grandi opererebbero ed opereranno molto meglio se sapranno adeguare la loro *governance* alla dimensione ed alla funzione che effettivamente hanno da anni.

In realtà, tutto questo non ha nulla a che vedere con questo provvedimento: è pura retorica, se andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Venendo poi al contesto europeo, perché dobbiamo ricordare che facciamo parte dell'Unione europea e dell'area dell'euro, non possiamo disconoscere quello che sta succedendo in Europa, il fatto che si è costituita un'Unione bancaria europea, c'è un meccanismo di vigilanza unico, che ci sono appunto banche sistemiche che sono in qualche modo vigilate ormai a livello europeo e ben sette di queste dieci banche popolari di cui parliamo

una misura che va completata e rafforzata e che c'è ancora molto da lavorare in questo campo: si tratta però di lavorare a Bruxelles e a Francoforte, non prendendocela solamente con alcune delle norme e dei criteri che abbiamo approvato insieme agli altri Paesi. È un dato di fatto che quello che le autorità di vigilanza europea in qualche modo ci segnalano è proprio l'allarme sul settore di queste dieci banche popolari, con riferimento

Questo ha un effetto importante: le esigenze di ricapitalizzazione sono più rilevanti per le banche popolari e lo saranno naturalmente e presumibilmente anche nel prossimo futuro. poi un problema di *governance* per quanto riguarda la capacità di provvista di nuovi capitali di questo sistema di banche. È un dato di fatto, tra l'altro già emerso, e ricordo a tutti che cosa è accaduto con gli ultimi *stress test* a livello europeo, con la faticosa rincorsa degli ultimi mesi per poter in qualche modo rientrare in quei parametri. Quello che si vuole fare, transitando queste banche nel modello delle società per azioni, è rafforzarle: in qualche maniera si vuole rafforzare la loro capacità di dotarsi della necessaria quantità di capitale.

sicuramente ci sarà anche il rischio di scalate ostili, com'è stato detto, ma non ci sono soluzioni definitive e ottimali. Vanno comunque giudicate positivamente le modifiche che sono state apportate alla Camera tra cui, com'è stato ricordato, il fatto di stabilire che i nuovi statuti potranno essere deliberati dalla stessa assemblea dei soci

è una misura che può in qualche modo aiutare a disincentivare le scalate ostili. Naturalmente è giusto dire che la nostra strategia non deve essere solo difensiva, ma anche offensiva, nel senso che bisogna accompagnare questo processo di trasformazione che in qualche maniera porterà al consolidamento del sistema delle banche popolari.

Sono affermazioni in libertà, che non si capisce su che cosa facciano poi perno e su che cosa si fondino. La verità è che, sullo sfondo dei grandi cambiamenti del sistema creditizio europeo ed internazionale, che ho menzionato all'inizio di questo mio breve intervento, credo si possa dire che questo provvedimento, insieme ad altri che naturalmente completeranno la ristrutturazione del sistema bancario e di intermediazione italiano mi riferisco allo sviluppo del credito non bancario, alle autoriforme delle banche di credito cooperativo, alla soluzione dei crediti deteriorati - potrà contribuire

mitico passato, ma quella di accettare le sfide che vengono dal contesto europeo ed internazionale, rispondendo positivamente attraverso misure che possano rafforzare questo nostro sistema. È per questi motivi che esprimo un giudizio positivo e sono quindi favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

intervengo pochi minuti per focalizzare alcuni punti di questo dibattito, che ho seguito molto attentamente. di ricordare il contesto internazionale ed europeo, perché lo ha fatto molto bene il collega Guerrieri Paleotti e che pure avevo sottolineato nella relazione iniziale.

sul sistema bancario in cui viviamo e in cui l'Italia e l'Europa sono immerse a pieno titolo,

e al credito locale, quindi alla maggiore capacità di legame con il territorio; l'altra, la soglia degli otto miliardi.

consentire una migliore messa in rete di tali realtà, diffuse sul territorio, che hanno certamente un legame territoriale, perché insistono su limiti territoriali definiti

Si tratta di banche che ormai hanno una dimensione nazionale, che svolgono una funzione che coinvolge mercati nazionali e sovranazionali, che hanno quindi una dimensione che non è più

Da questo punto di vista, anche quest'aspetto non appare di grande rilevanza. In effetti, differenza tra la soglia degli 8 miliardi e quella dei 30 interesserebbe solamente tre banche,

pertanto davvero a lasciare da parte tutta una serie di considerazioni che trovo sbagliate. Si tratta quindi di una riforma che, sotto tale profilo, costituisce un elemento assolutamente positivo, che dà la giusta veste giuridica a banche di dimensioni che si devono confrontare con una realtà come quella che abbiamo indicato all'inizio della discussione in corso e che è stata molto ben ricordata dal collega Guerrieri Paleotti.

la critica, se non l'intera discussione generale, si è concentrata sulla parte del provvedimento dedicata alle banche popolari, su

registrare un sostanziale consenso, non solo della maggioranza, ma anche di parte dell'opposizione, quantomeno sul resto del provvedimento. I colleghi Castaldi e Martelli hanno espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul sistema delle *start up* innovative. Il collega Martelli ha contestato alla alla società per la patrimonializzazione e la ristrutturazione di imprese in crisi il fatto di essere uno strumento per salvare l'ILVA di Taranto. Questa, dal nostro punto di vista, non è

senatrice Pelino, che ha contestato essenzialmente alle agevolazioni previste per le piccole e medie imprese innovative la loro portata limitata ed il fatto di essere funzionali soltanto agli investimenti sulla ricerca e sullo sviluppo, nonché di rappresentare sostanzialmente semplificazioni di carattere formale, è agevole obiettare che, se così fosse, sarebbe già tanto. Il sostegno alla ricerca è infatti condizione imprescindibile per l'innovazione e lo sviluppo, mentre la semplificazione degli adempimenti formali è proprio quello di cui ha bisogno il nostro sistema delle delle piccole e medie imprese, per liberare le proprie energie. Il fatto è che così non è e che in questo provvedimento per le piccole e medie imprese innovative vi è molto di più: le agevolazioni fiscali per gli amministratori, per il personale, per i collaboratori, per chi investe nel capitale sociale di queste società; l'accesso semplificato, diretto

la possibilità di reperire capitale di rischio dal mercato per il tramite di portali *on line*; insomma, c'è molto altro.

Il decreto-legge è molto articolato e contiene materie valide ai fini della crescita e dello sviluppo del Paese, come hanno opportunamente sottolineato questa mattina la senatrice Fabbri e poc'anzi il relatore cito soltanto la portabilità dei conti correnti, gli strumenti più efficaci a sostegno dell'internazionalizzazione delle nostre imprese e del sistema economico italiano, le *start up* innovative, il potenziamento del fondo per le piccole e medie imprese. Invito a non sottovalutare tutte queste parti, perché sono davvero utili e su molte di esse si è registrato un consenso ampio oltre la maggioranza. Ma veniamo al merito dell'articolo 1. Sono note e discusse le ragioni che hanno portato il Governo a prendere la decisione di intervenire su questa materia. Tutti, da qualsiasi parte, anche coloro che hanno criticato aspramente il provvedimento, hanno riconosciuto la necessità e l'importanza di una riforma. Ebbene, visti anche i solleciti da parte delle autorità bancarie europee e nazionali e dopo gli esami fatti dalla banca europea

per non lasciarla priva di una struttura di riordino di un settore così strategico per il nostro Paese. La ragione che ci ha portato ad intervenire è molto semplice ed è stata ricordata in molti interventi, dalla senatrice Ricchiuti stamattina e da molti altri: distinguere tra la vera natura popolare, mutualistica e territoriale - sottolineo territoriale del sistema bancario popolare e la natura commerciale *tout court* che, all'interno dello stesso sistema, è prevalsa nelle banche, soprattutto le più grandi.

Non demonizzo questo, ma certamente non me la sento dire che questo è l'esempio clamoroso di democrazia economica. Non c'è alcun attacco alla democrazia economica e alla natura stessa delle banche popolari. La riprova qual è? Si interviene solo su 10, le più grandi, su 70. È stato rilevato che le altre 60 banche sono piccole, ma non sono toccate né nella natura, né nella *governance* e il fatto che siano piccole in un numero così rilevante, forse ha anche qualche attinenza con la loro prevalente mutualità In secondo luogo, le fondazioni bancarie non sono toccate. In questi giorni è stato fatto un accordo tra il Governo e le fondazioni bancarie per un sistema di auto regolamentazione. Ma perché in questo decreto-legge non sono presenti le banche di credito cooperativo? Ce lo chiediamo? Se ci fosse un attacco così viscerale alla democrazia economica, dovrebbero stare dentro un provvedimento così pesante, pesante, come viene denunciato. No, sono fuori, perché è in atto con loro (innanzitutto da loro stessi e con loro) un processo di autoriforma importante ed interessante. Quindi, escludo qualsiasi attacco alla democrazia economica; anzi, penso che stiamo tutelando le vere popolari. E poi c'è la soglia degli 8 miliardi che va in questa direzione. Ci potevano essere altri criteri, che sono stati discussi a lungo, anche nel dibattito alla Camera. alla Camera. La vigilanza si colloca a 30 miliardi. La valutazione che ha fatto il Governo è che questa soglia, per il sistema delle popolari italiane, è troppo elevata rispetto alla comprensione del cambiamento di natura mutualistica. C'è il criterio delle quotate, certamente, ma - attenzione - ci sono alcune quotate che che non sono SpA, perché sono piccole. Se noi avessimo detto che *a priori* le quotate diventano SpA, le avremmo obbligate tutte indipendentemente dalla loro dimensione. Alla Camera si è anche discusso quelle che hanno delle SpA nei gruppi. Tutto questo è stato valutato, ma le controindicazioni che ho ora brevissimamente citato hanno portato a scegliere la linea della soglia. Stamattina la senatrice Pelino ci ha chiesto di non scartare una riflessione futura su questi temi. Bene, credo che sia assolutamente ragionevole dire che non sono temi accantonati. Noi oggi scegliamo una soluzione,

posso dire con molta chiarezza che tale soluzione può non essere condivisa, ma non si dica, per favore, che non ne è stato mai spiegato il perché. È stato spiegato più volte, in pubblico, in Aula, in Commissione, alla Camera. Quindi, è molto chiaro il perché. La valutazione che abbiamo fatto ci ha portato ad una soglia che si colloca - come dice la relazione che introduce il decreto-legge - ad un punto intermedio tra la quotazione massima e la quotazione minima, considerando quindi che quella poteva essere una valutazione di soglia che consente di affermare, anche valutando la distribuzione territoriale, che le banche che stanno sopra hanno in qualche modo superato la loro natura mutualistica.

che un'anomala situazione che dovesse verificarsi (cioè una contemporaneità di recessi, soprattutto in fase di trasformazione) finirebbe per penalizzare la capitalizzazione della banca stessa. Che la prova sia solo questo e non altro è data dal fatto - ad esempio - che, su un caso clamoroso dove non esiste questo rischio (cioè in caso di morte del socio), il divieto di recesso è stato tolto. è stato tolto. In quel caso, infatti, è del tutto evidente che non c'è alcuna attinenza tra il fatto in sé e l'effetto che potrebbe esserci sulla capitalizzazione delle banche. Mentre invece la prudenza, soprattutto in questa fase di trasformazione, vuole proprio che si eviti che una coincidenza di recessi provochi un danno alle stesse popolari È chiaro che tutto questo si è sviluppato, ma poi alla fine - come ha ricordato anche il presidente Mucchetti - la questione vera si è rivelata essere la scalabilità delle banche, soprattutto rispetto al rischio della

Da questa condivisione deriva l'accoglimento della proposta di limitare l'esercizio di voto, con la scelta adottata del 5

Quindi, noi consentiamo un vantaggio alle banche popolari che si trasformano: possono, cioè, adottare il limite di voto con una maggioranza più facile di quella altrimenti necessaria.

le allieve, gli allievi e i docenti dell'Istituto «Salvatore Quasimodo» di Ragusa, che seguono i nostri lavori.

spero che venga per ritirare questo provvedimento e, per tutte le buone ragioni che sono state illustrate, per presentare un disegno presentare un disegno di legge che possa validamente affrontare la questione delle banche, delle banche popolari, delle banche di credito cooperativo. si autodenuncia persino come non avente i presupposti di costituzionalità di straordinaria necessità e urgenza, perché nella sua premessa dice che la straordinaria necessità e urgenza sta nell'avviare il processo di adeguamento al sistema bancario e agli indirizzi europei. Da nessuna parte, negli indirizzi europei, ci sono i limiti che vengono proposti in questo decreto-legge, che è già in vigore da parecchie settimane e interviene su diritti di proprietà, sul diritto al sostegno alla cooperazione e sul diritto alla libertà d'impresa. aspetti sono intervenute e sono già in vigore da settimane norme palesemente contrarie a parecchi articoli della Costituzione. Ci sono mille ragioni per dire: fermiamoci facciamo una procedura normale; applichiamo veramente gli indirizzi europei; guardiamo agli esempi degli altri Paesi. Se si parla con gli imprenditori, quelli che hanno la possibilità di creare occupazione, tranne quando lo Stato decide di assumere decine di migliaia di persone, magari senza concorso e andando anche in questo caso contro la Costituzione - in genere l'occupazione viene prodotta dalle imprese - si comprende che le imprese hanno alcuni nemici mortali

gli intoppi burocratici, una macchina fatta apposta per scoraggiare chi vuole fare le cose, specialmente se vuole farle per bene. Il terzo nemico, forse il più importante - non siamo, però, solo noi a parlare con gli imprenditori e con possibili investitori è l'impossibilità di avere credito dalle banche. Chi in questi anni è riuscito comunque a garantire delle linee di credito, è venuto incontro alla piccola e media impresa ed alle esigenze del territorio? Le banche popolari. Ebbene, cosa fa questo provvedimento? Le prende d'assalto e, e, cambiando loro natura, le fa diventare come le altre: quelle stesse altre che, per varie ragioni, negli ultimi anni non hanno garantito questo fondamentale elemento alla nostra economia. Il sottosegretario Baretta, illustrando alcuni elementi realmente positivi, che forse sono contenuti in questo provvedimento, ci ha detto

ci porta come esempio la più grande banca singola, che comunque sarebbe effettivamente al di sopra dei limiti esistenti in Germania. Ma le *Volksbank* e le *Landesbank* sono state preservate dal Governo tedesco negli interessi del popolo e delle imprese tedesche. Ci vorrebbe anche un Governo italiano che garantisse gli interessi delle imprese e dei cittadini italiani.

sono stati ripartiti 20 minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto. La chiama avrà pertanto inizio attorno alle ore 19,30.

Signor Presidente, con il decreto-legge sulle popolari il Governo ha deciso che le banche a voto capitario, superiori alla dimensione di 8 miliardi di euro di attivo, sono inadatte a sopravvivere sui mercati finanziari globali e a contribuire al bene comune. Peccato che il resto del mondo non la pensi allo stesso modo. Non la pensa così l'Europa, perché le prime 50 banche a voto capitario nell'Unione europea hanno una dimensione media superiore ai 120 miliardi di euro di attivo e, quindi, ben oltre la soglia degli 8 miliardi di euro, che per il nostro Governo rappresenta il confine tra il possibile e l'impossibile, tra il bene e il male. Non ce lo chiede neanche la Merkel, perché la stessa ha deciso di ricapitalizzare pubblicamente le proprie grandi banche popolari, le *Volksbank*, ritenendole un pilastro fondamentale dell'economia sociale di mercato. Le nostre non hanno bisogno di ricapitalizzazioni pubbliche, ma le chiudiamo, mentre usiamo soldi dei contribuenti per cercare di far ripartire alcune esperienze fallimentari di banche SpA, come quella del Monte dei Paschi. I colleghi olandesi, tedeschi, austriaci, francesi e finlandesi, le cui economie beneficiano dell'apporto di grandi banche a voto capitario, si chiedono stupefatti cosa stia accadendo in Italia. Sono perplessi gli amici canadesi, che hanno probabilmente il miglior sistema finanziario del mondo, non toccato dalla crisi, con un modello di banca a voto capitario che ha conquistato più del 40 per cento Dovrebbe essere proprio il mercato, i cittadini consumatori e risparmiatori, in normali condizioni di libertà e democrazia, a decidere in quale modello di banca vogliono investire i propri risparmi. Da noi invece è il Governo, a differenza di quanto deciso negli altri maggiori Paesi ad alto reddito, a limitare con un editto questa nostra libertà. Peccato ancora che dati nazionali ed internazionali ci ricordano che, negli ultimi anni, le banche a voto capitario, e in particolare le popolari, hanno erogato, in proporzione al loro attivo, significativamente più credito ad imprese e famiglie delle banche SpA, laddove queste ultime, stressando il principio della massimizzazione dell'utile, non hanno oggi più interesse a dedicarsi ad un'attività a basso rendimento e ad alto rischio, come far credito, in un mercato altamente competitivo. Il risultato di questo decreto-legge sarà, dunque, quello di inaridire una fonte importante di credito ad imprese e famiglie e di lasciarci soli con un modello di banca che, per sua natura, cerca di vendere di tutto allo Non è un caso che, di fronte a questa radicale contraddizione tra ricerca del massimo profitto

Non ce n'è bisogno, basterebbe molto meno, ovvero lasciare in vita e rinforzare il modello di banca a voto capitario, non massimizzatrice di profitto, e muovere verso la separazione tra banche d'affari e banche commerciali, come stanno facendo le principali economie ad alto reddito mondiali. banche popolari noi andiamo, invece, contro mano e - come ha detto un giornalista de «la Repubblica», non senza ironia - come possiamo aspettarci che le pratiche di fido degli artigiani veneti, che verranno esaminate in qualche lontana capitale oltreoceano, vengano preferite, con i loro miseri rendimenti (miseri per la banca, ovviamente), a qualche operazione finanziaria di *trading*, assolutamente più redditizia? I rapporti di molte organizzazioni internazionali a favore della biodiversità bancaria, gravemente lesa da questa decisione, confermano che non esiste alcuna motivazione economica o giuridica a supporto di tale scelta. La biodiversità è fondamentale perché tipologie di crisi diverse colpiscono in modo selettivo diversi modelli di banca, e avere diversità e ricchezza rende i sistemi più resilienti. Le banche a voto capitario, come dimostrano gli studi economici, hanno minore volatilità degli utili e maggiore intensità di credito sul totale dell'attivo; averne di meno indebolirà il nostro sistema finanziario, esponendolo molto di più ai rischi di nuove gravi crisi finanziarie, lasciandoci con banche pericolosamente esposte verso il *trading* speculativo e senza la protezione - come in molti altri Paesi - della separazione tra banca commerciale e banca d'affari. Vivremo il paradosso e la beffa di ridurre la capacità del nostro sistema bancario di finanziare famiglie e imprese, proprio nel momento in cui la Banca centrale europea ci inonda di liquidità, sperando che essa finisca per alimentare il credito. Le dieci banche colpite hanno passato gli *stress test* meglio della media del settore e hanno dimostrato di poter raccogliere capitale rapidamente nei momenti di bisogno, perché gli investitori guardano alla qualità di una banca e non alla possibilità di ottenerne il controllo. Le banche popolari, come ogni modello di banca, hanno i loro pregi e i loro limiti e, per curare questi limiti, esistevano ricette molto più opportune, relative alle regole di voto, al ricambio delle classi dirigenti, ai fondi di ricapitalizzazione secondo modalità già adottate per il sistema delle Ma soprattutto, la presenza di un limite alla libertà di iniziativa economica è un assunto giuridico, che sarà spazzato via dal primo ricorso alla Corte costituzionale avviato dai soci delle vecchie banche a voto capitario. [**Presidenza del vice presidente come confermato da quattro illustri pareri di costituzionalisti (Ainis, Flick, Mirabelli e Imposimato), che hanno sottolineato come il *golpe* sulle banche popolari violi sette articoli della Costituzione - non uno, ma sette soprattutto il 45, che dichiara che l'Italia sostiene e promuove la crescita della forma cooperativa in economia. Quando il ricorso avverrà e la Corte costituzionale darà ragione ai ricorrenti, la sciagurata decisione di oggi si rivelerà un *boomerang* per lo stesso Governo, producendo ulteriore confusione, *caos* e ulteriori strascichi tra i soci delle banche popolari. È quello che dobbiamo assolutamente evitare e che oggi potremmo evitare, se prendessimo la saggia decisione di accantonare la conversione La storia renderà ragione e ci consentirà di capire pienamente quello che è successo in questi mesi. Per ora ci resta, purtroppo, lo squallore della cronaca. Abbiamo ancora un'ultima occasione per non essere complici,

Presidente, siamo nella fase della discussione generale sulla questione di fiducia e, quindi, vale la pena estendere un po' il ragionamento, anche se il tempo concesso è molto breve.

Attorno a questo tema, tutti quanti noi ci saremmo aspettati una discussione adeguata da parte del Parlamento, nel rapporto e nel confronto con le parti sociali, con il sistema delle imprese: un dibattito che è nella responsabilità del Governo attivare, sostenere e portare a sintesi per migliorare la qualità delle

non discussa, ma annunciata ed anche coerentemente portata avanti, nella quale la condizione necessaria è individuata nella assenza del dibattito, nella cancellazione del confronto, nella riduzione degli spazi e degli ambiti di intervento da parte sia del sistema più ampio delle imprese, che non si chiude in Confindustria, che del sistema del sistema sociale, delle organizzazioni sindacali e soprattutto da parte del Parlamento. Signor Presidente, penso che quello che dobbiamo assolutamente è un dovere che riguarda anche il suo ufficio, cioè il governo di questa Camera, perché non fa bene al Paese e non produce effetti positivi, la mortificazione della discussione, la mortificazione di una ricerca delle soluzioni, che veda partecipi tutti gli interessati, che sono i cittadini e le loro rappresentanze, ma che sono anche le organizzazioni sociali ed il sistema delle imprese che - come dicevo - non si riduce ai soli aderenti alla Confindustria. Purtroppo, questo non sta avvenendo. Questo decreto-legge, con l'ennesima fiducia su una questione che attiene all'economia del Paese, lo dimostra: arriva dopo 50 giorni, pieno di vizi di natura costituzionale; incamera un voto politico sulla sua costituzionalità; dopo di che va a discussione sterile, ad un esame della Commissione solamente formale ed, infine, viene posta la fiducia. Andando avanti così, è meglio che il Parlamento rinunci

luogo, perché sono riusciti in mezza giornata a portare a casa il provvedimento. Con cinque minuti di dichiarazioni di voto si chiude infatti baracca e burattini, perché oggi il decreto-legge scade e lo si deve portare a casa. Complimenti a Renzi e complimenti alla sua maggioranza,

tanto le banche di credito cooperativo quanto quelle popolari sono quelle che hanno resistito alle turbolenze ultime del mondo finanziario nel migliore dei modi e c'è un perché. le banche popolari hanno maturato meno sofferenze? Per il semplice motivo che hanno una struttura con a capo dei direttori che conoscono il territorio:

Il problema è uno ed è semplice: chi ha bisogno di denaro e non lo trova in banca non ha una seconda via, non c'è il sistema pubblico o privato, ma si deve rivolgere ad un sistema illegale!

sulla questione di fiducia, al termine di un importante dibattito che, pur nei tempi ristretti, il Senato ha saputo e ha voluto svolgere su un tema così importante.

netta divisione che si sta evidenziando in quest'Aula tra i sostenitori della democrazia economica e quelli della finanziarizzazione dell'economia. Cala la maschera sul fatto che abbiamo assistito in questi ultimi anni - da quella crisi finanziaria che presto si è trasferita sull'economia reale e che è arrivata a picchiare duro anche da noi al presunto atteggiamento di impotenza da parte di Governi e Parlamenti, che in realtà nasconde solo l'incapacità a capire e a comprendere che nella storia europea e del nostro Paese c'erano e ci sono, forse ancora per soli diciotto mesi, i capisaldi della possibile reazione a questa drammatica crisi che, all'interno della globalizzazione, accompagna come un canto di morte, attraverso gli eccessi della finanza, la sorte dell'economia reale. Mi riferisco all'economia del lavoro, a quella che

proprietà legittima di persone che, con un modello cooperativo, si sono associate, organizzate e svolgono un importante ruolo nel sistema economico: assistere l'economia attraverso la

oltre all'esproprio, il trasferimento di ricchezza, che dalle banche dei territori passerà rapidamente - come ho già detto prima - a intermediari finanziari o a banche di affari che, alla City di Londra piuttosto che a Wall Street, decideranno come sarà fatto il credito nel nostro Paese e su chi investire per privilegiare un tipo di economia piuttosto che un'altra. Per esempio, sarà ancora l'economia della manifattura o sarà solo l'economia dei servizi ad essere

costituzionalmente previsto, finalizzato alla tutela del risparmio? Stiamo tutelando il risparmio degli italiani? No, con questo decreto stiamo regalando il risparmio degli italiani a grandi investitori stranieri che ne faranno certo un buon uso, di sicuro non un buon uso per il nostro Paese. Gettino pure la maschera coloro che ancora ci raccontano che questo decreto-legge serve a consolidare il sistema bancario italiano. No, questo decreto, come già avvenuto

anche all'interno della crisi finanziaria scatenatasi negli ultimi anni, su banche che non avevano bisogno di alcun consolidamento. Avevano solo la necessità di di essere rispettate nella loro prerogativa costituzionale. Qualcun altro, invece, aveva bisogno che le banche popolari venissero costrette a vendere le loro azioni per essere acquistate a pochi soldi e quindi svendute sul mercato finanziario internazionale.

il Governo fosse in Aula, non soltanto con la persona del sottosegretario Pizzetti, sempre ottimamente presente, ma almeno con chi è competente per materia. Onorevoli colleghi, vorrei solo per un attimo estraniarmi dai rilievi tecnici del voto capitario piuttosto che del tetto degli otto miliardi e ragionare di qualcosa della quale fatico a capire se abbia ancora diritto di cittadinanza in quest'Aula. Vorrei, cioè, parlare di politica; e poco importa se si tratti di politica economica o di politica *tout court*. Dirò allora che "il modo ancor c'offende": provo ad usare la lingua del più illustre dei toscani, giusto a verificare se mi riesce di sintonizzarmi con un Governo che fatica a comprendere le ragioni della stragrande maggioranza degli italiani, con buona pace di tutti quei battitori di grancassa che allignano in ogni settore della comunicazione, i più proni dei quali siedono comodamente in casa di mamma RAI. il modo ancor c'offende, perché questa nuova riforma ripropone pari pari un problema di metodo che è ormai diventato il problema, quello cioè dei rapporti fra il Governo ed il Parlamento. Anche oggi, come ieri, vale la pena sottolineare che questo Parlamento non è contro le riforme: eravamo e siamo d'accordo sul superamento del bicameralismo perfetto, così come eravamo e siamo d'accordo sulla riforma del sistema della *governance* delle banche popolari. Non siamo però più disponibili ai *Diktat* di Palazzo Chigi sul modello prendere o lasciare. Ha voglia il Presidente del Consiglio di cinguettare della pigrizia dei professori che parlano di deriva autoritaria, ma tant'è: se si parla per fatti concludenti e li si mette uno di fila all'altro, appare chiaro che questo Governo ci sta conducendo verso una plutocrazia fatta dai Perotti al servizio delle grandi imprese che non amano la libera concorrenza, con a capo un disinvolto ibrido, metà Primo Ministro, metà segretario di partito unico, come le primarie di Agrigento ci insegnano. È così. stata la riforma delle Province, con cui l'unica cosa che è stata abolita sono le elezioni, come a dire: «Questi cittadini elettori sono un fastidio, facciamo in modo che siano direttamente i partiti a scegliere chi amministrerà le Province», che quindi esistono e continueranno senza controllo elettorale ad amministrare risorse pubbliche, con Renzi sempre a dirigere il partito-Stato. Vi è poi stata la riforma della Costituzione, nella quale, oltre a ridurre - anzi, direi annullare - gli spazi di democrazia,

la riforma elettorale, contrabbandata con lo *slogan* «perché gli italiani devono sapere subito chi ha vinto», quando invece la traduzione letterale del Renzi-pensiero è: «perché gli italiani devono sapere subito che ho già vinto». Tralasciando altro, arriviamo alla riforma delle banche popolari, sempre con uno *slogan* tipicamente populistico: «Ci sono tantissimi banchieri e pochissimo credito alle famiglie e alle piccole e medie imprese». Anche qui, la traduzione è semplice: «Nelle banche popolari ci sono i risparmi degli italiani, il bottino è buono, prendiamoceli e decidiamo noi come investirli». Ho apprezzato molto l'intervento del senatore Mucchetti, che con dovizia di particolari ha sbugiardato la maggior parte dei presupposti che motivano questa riforma. Su un solo punto dissento, là dove, nell'adombrare circostanze poco chiare e commendevoli verso questa riforma, suggerisce di non entrare nel territorio del sospetto. Senatore Mucchetti, noi nel territorio del sospetto dobbiamo entrarci, anzi: abbiamo l'obbligo d'indagare e sapere, perché, se non lo facciamo, ci ritroviamo poi con gli Incalza e gli Odevaine,

allora chiaramente e chiediamocelo: l'asticella degli otto miliardi di attivo, anziché i 30 previsti dalla normativa europea, serve a salvare la Banca popolare dell'Etruria? Sul malcostume normativo della decretazione d'urgenza, che ormai caratterizza questa legislatura, con decreti-legge che non hanno il minimo requisito della necessità e dell'urgenza, come Costituzione imporrebbe e lo sottolineo verso il neoeletto Presidente della Repubblica - la riforma delle popolari serve forse a trovare una soluzione per il Monte dei Paschi di Siena? Ancora: si dice di una riforma che aspettiamo da vent'anni. A me pare strano, forse mi sono informato da qualche altra parte, però le banche popolari sono state oggetto di una riforma - leggendola con la stessa lente del Governo - nel "lontanissimo" 17 dicembre 2012, con la Cosa diceva quella legge? Introduceva rilevanti aperture al peso del capitale, ha innalzato i limiti al possesso azionario raddoppiandoli, ha innalzato il limite al possesso per i soggetti risultanti da operazioni di aggregazione, ha ha subordinato i diritti amministrativi, tra cui il voto al possesso di un pacchetto minimo di azioni, ha previsto quote riferite al capitale per l'esercizio dei diritti sociali. Concludendo, signor Presidente, la riforma delle banche popolari è stata caratterizzata da un'ampia e quanto mai oscura vicenda, legata a fughe di notizie e possibili attività di *insider trading,* su cui la CONSOB ha già avviato un'indagine un'indagine subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto-legge. Il Governo e la maggioranza, noncuranti delle note criticità contenute nel decreto-legge, intendono approvare un atto legislativo profondamente illiberale, perché limita la libertà di impresa. Ma c'è qualcosa di più. È stato violato l'articolo 3 della Costituzione, tra banche e cooperative che sono costrette ad essere trasformate in SpA ed altre, invece, che non lo sono. Le norme contenute riguardano tutte quelle imprese che superano, come abbiamo detto, gli 8 miliardi di attivo, e non si capisce perché la stessa norma non sia stata equiparata a quanto prevede la legislazione europea. C'è poi una questione delicatissima, quella del diritto di recesso: il decreto-legge interviene sul diritto di recesso per evitare che il rimborso delle azioni possa riflettersi negativamente sulla computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Si attribuisce alla Banca d'Italia una potestà generale in relazione a tutte le ipotesi di recesso. Ma ancora: il decreto, oltre alle ripercussioni sulle economie locali, andrà a distruggere il rapporto che dura ormai da tantissimi anni tra le banche popolari, le famiglie e le piccole e medie imprese. Da ultimo, una sorta di *coup de théâtre*, signor Presidente: l'articolo l'articolo 7 resuscita come d'incanto la GEPI e le partecipazioni statali. Qui il miracolo di Renzi verrà compiuto: avremo più Stato e più società per azioni. Penso ce ne sia abbastanza per annunciare il mio voto contrario e quello del mio Gruppo, lasciando comunque una diversa

Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto prego il presidente Calderoli di voler estendere al presidente Grasso le congratulazioni da parte del nostro Gruppo perché in sei giorni, da

una tradizione del Governo Renzi ispirata dall'altro tristemente noto Governo, quello di Monti, un Governo non legittimato dal popolo. Decreto-legge e fiducia: il classico andazzo di questi Governi che si sono succeduti. Questa importante riforma, che dovrebbe mettere mano a centocinquant'anni di storia del nostro Paese - le banche popolari - avrebbe dovuto avere, a nostro giudizio, un *iter* parlamentare degno di quella storia e del Parlamento stesso. C'era tutto il tempo per affrontare la riforma con un *iter* parlamentare ordinario, con il contributo del Parlamento, ma anche accogliendo le legittime istanze delle parti sociali coinvolte da questa riforma. Niente. Chiusura pressoché totale. Per cui, presidente Renzi, se la voti lei questa fiducia, l'ennesima fiducia. Noi non parteciperemo a questa commedia; la voti lei, con i suoi servi e con i suoi camerieri! *(LN-Aut)*. Ma su questa riforma non pesa solo l'arroganza del Governo; c'è pure una questione morale e forse anche giudiziaria, sulla quale abbiamo chiesto e continueremo a chiedere chiarimenti. Mi riferisco, se qualcuno finge di non capire, alla Banca popolare dell'Etruria, della quale il ministro per le riforme Maria Elena Boschi è azionista,

Un caso? Ce lo sapranno dire la procura di Roma, che sta indagando, e la CONSOB, impegnata a ricostruire gli scambi di quei giorni. caso, presidente Renzi, ministro Boschi, ci saremmo aspettati da parte vostra la stessa chiarezza e determinazione usate in occasione dei problemi che hanno portato alle dimissioni del ministro Cancellieri nel 2013, per - cito - rapporti poco chiari fra il Ministro e finanzieri/imprenditori. Sono parole del Primo Ministro. Sempre il Primo Ministro affermava che si trattava di una questione di prestigio delle istituzioni e di credibilità delle riforme. Sempre lei, presidente Renzi, sosteneva che qualsiasi posizione sulla riforma della giustizia avrebbe scontato un giudizio diffidente di larga parte degli italiani; e aggiungeva (sempre parole sue): «Il PD deve fare una solenne promessa: che di fronte alle regole del mondo dell'economia la politica non è più succube degli interessi delle famiglie e degli amici degli amici, ma prova a fare un percorso in cui la legge è uguale per tutti». E bravo il vostro Matteo, che a gran voce chiese le dimissioni del ministro Cancellieri! Opportunità politica? Chi lo sa. Non vogliamo Non vogliamo allora chiedere anche le dimissioni del ministro Boschi per opportunità politica? Oggi probabilmente questo principio non vale più. forse scordavo che in quel tempo Enrico Letta stava ancora sereno, o non stava ancora sereno. Quanto a lei, ministro Boschi, che rispetto al novembre 2013 - mi creda - ci sembra un'altra persona, nella stessa occasione, sempre nella lotta per il controllo della segreteria del PD, sentenziava candidamente, con il sorriso sulle labbra che il ministro Cancellieri doveva dimettersi, aggiungendo: «Non pare ci siano profili di illegittimità nella sua condotta, ha dato l'idea profondamente sbagliata di un sistema in cui solo se conosci qualcuno riesci a vedere tutelati i tuoi diritti». E io aggiungerei: anche i tuoi interessi.

pare che non ci siano profili di illegittimità nella sua condotta. Pare, ma, sotto l'aspetto morale, ce n'è a sufficienza. Stia serena e speriamo che la CONSOB e la procura di Roma facciano il proprio lavoro. Archiviata temporaneamente la parte morale che vi riguarda direttamente, veniamo al vostro decreto-legge. Anche qui di morale ce n'é ben poca. La riforma delle banche popolari è incostituzionale, discriminatoria, superficiale e crea danni incalcolabili, oltre a mettere a rischio 20.000 posti di lavoro (dato Assopopolari). Il Governo svende per decreto oltre centocinquant'anni di storia economica del Paese e sottrae ai territori in maniera incondizionata la ricchezza che hanno generato, gettando in pasto ai grandi interessi speculativi istituti solidi che hanno contributo alla crescita economica del Paese, oltre al fatto di garantire il credito in questo momento di profonda crisi. Noi abbiamo una visione diversa da quella del Governo: per noi le banche popolari non sono un'anomalia da superare, per noi le nostre banche sono un valore da tutelare. Ma allora perché tanta fretta? Ce lo chiede l'Europa; ce lo chiede *frau* Merkel, ancora una volta. Chiedete allora alla Merkel cosa ne pensa del *crack* che proprio in questi giorni rischia di far fallire in Austria, oltre alla alla banca Hypo Alpe Adria, con un buco di oltre 10 miliardi di euro, un'intera regione, la Carinzia, con il rischio di produrre un effetto domino in tutta Europa. È uno scandalo di cui pochi parlano e che è già stato battezzato come il caso Lehman Brothers d'Europa; e voi cosa fate? Con questo clima di incertezza e instabilità della *governance* bancaria offrite le nostre banche su un piatto d'argento ai grandi speculatori internazionali, gente senza scrupoli e senza morale che azzanneranno le nostre banche, le spolperanno fino all'osso per il raggiungimento dei propri profitti, per poi liberarsene senza troppi scrupoli, alla faccia della nostra storia, della nostra economia e del nostro Paese. Siete degli irresponsabili! I banditi, come ricordavo prima, della tristemente nota vicenda Lehman Brothers hanno pregiudicato il sistema finanziario globale, con conseguenze che, ancora adesso, anche nel anche nel nostro Paese, i cittadini stanno pagando. Questi finanzieri, che sarebbe meglio definire delinquenti dell'alta finanza, probabilmente hanno complici nel nostro Paese, già pronti ad assecondare la loro ingordigia pronti, anche loro come voi, ad assecondare i grandi interessi speculativi internazionali. State rappresentando un bel quadretto. Tra la vostra moralità e quella di coloro ai quali offrite le nostre banche fate proprio un bel quadretto. Mi sembra «L'urlo» di Munch.

e si fa per dire - parleremo tedesco, se ci andrà male, parleremo cinese. Ma la cosa che ci angoscia di più, tanto per restare in tema, è l'immagine che questo Governo vuole consegnare alla storia del nostro Paese, continuando ad assecondare il volere dell'Europa, la finanza creativa e l'economia di carta. È un'immagine già vista: quella dei dipendenti della Lehman Brothers con lo sguardo basso, gli occhi lucidi e gli scatoloni in mano. Questo volete consegnare al nostro Paese!

non ha molto senso. Come faceva saggiamente notare il collega Carraro tempo fa, diventa la fiera delle vanità e basta. Questo è un provvedimento che contiene molti elementi, alcuni anche abbastanza interessanti, se avessimo avuto il tempo di approfondirli. In esso, però, di fatto il piatto forte

Un provvedimento per il quale, ad ogni motivazione addotta dal Governo, se ne trova una contraria che smonta la teoria, a partire dalla necessità e urgenza che avrebbero portato all'utilizzo dello strumento del decreto, urgenza che si scontra con le tempistiche contenute nel decreto stesso. Ricordiamo che ci sarà l'emanazione delle norme operative da parte di Bankitalia e, quindi, diciotto mesi per adeguarsi. La giustificazione data in Commissione su questo tema, e ribadita anche in questa Aula, a me appare paradossale: l'urgenza era nell'emanare il provvedimento. C'era l'urgenza per l'urgenza. Ma io mi chiedo se l'urgenza sia quella di consentire a qualcuno una bella speculazione in Borsa. Viste le tempistiche cui accennavo, quelle previste dal decreto, concedere anche solo poche settimane in più a questo ramo del Parlamento che, è bene ricordarlo, ormai da mesi sta affrontando una importante indagine conoscitiva proprio sul sistema bancario italiano, avrebbe sicuramente aggiunto valore al provvedimento stesso, ne avrebbe sanato le criticità trasversalmente riconosciute ed avrebbe evitato di svilire per l'ennesima volta l'attività di questo Senato che si ostina ad esistere e lavorare. Ma forse questo è proprio un desiderato effetto collaterale del modo di agire di questo Governo: evidenziare l'inutilità di questa istituzione e di quanti in essa operano. Un'urgenza, dicevo, che non deriva dalle pressioni di quell'Europa con cui spesso ci si riempie la bocca. Di stroncare le popolari non ce lo chiede l'Europa, tantomeno il resto del mondo. Basta vedere come si comportano Francia e Germania nei confronti delle proprie banche popolari! Queste sono considerate un patrimonio e una ricchezza del sistema bancario e non un peso da sopprimere o smantellare. Senza dimenticare l'esempio canadese, con la Cassa popolare Desjardins che, come ricordava la collega Bonfrisco, Bloomberg ha definito la seconda banca più solida del mondo. E allora chi ce lo chiede?

Devo dire che non ricordo quando la Banca d'Italia abbia caldeggiato la trasformazione dei gruppi bancari Montepaschi e Carige in qualcos'altro che non fosse una SpA, pure considerando le note vicende che le hanno coinvolte. Ricordo, invece, che lo Stato italiano - quindi indirettamente i cittadini italiani - ha dovuto tirar fuori qualche soldino (in prestito, per carità) per salvare il gruppo Montepaschi, non questa o quella banca popolare. Incredibilmente ha urgenza anche l'Autorità sulla concorrenza, che auspica il concretizzarsi di un provvedimento che con la concorrenza fa proprio a cazzotti! Si è parlato in maniera dogmatica dell'assioma «troppi banchieri, poco credito»; peccato sia smentito dai dati (dati Bankscope, la maggiore banca dati mondiale disponibile sui temi bancari), che mostrano come, specialmente durante la crisi, sono le popolari ad avere mantenuto il più alto rapporto tra attivo e credito e ad avere l'offerta creditizia meno prociclica! Si è parlato di autoreferenzialità degli organi di amministrazione delle popolari e credo che sarebbe stato ragionevole, anche per le popolari stesse, avviare un percorso che aiutasse a superare in maniera compartecipata le asperità che sotto alcuni aspetti possono condizionarne in maniera negativa la *governance*, in modo da rendere il sistema delle popolari più moderno e rispondente all'attuale assetto del mercato del credito. Si è scelta, invece, la solita strada dell'atto di forza che, purtroppo, ricalca altri episodi di questa legislatura. Si è parlato di maggiore rischiosità delle banche popolari, collegando il fattore rischio al voto capitario, capitario, in aperto contrasto con un'ampia letteratura bancaria che non evidenzia alcun tipo di legame tra i due fattori, chiarendo invece che la maggiore o minore rischiosità di una banca deriva da tutt'altro: diversificazione del portafoglio, volatilità degli utili, facilità di raccolta fondi, solo per fare qualche esempio. Non solo, se facciamo un discorso di rischio sistemico, richiamo l'attenzione sull'importanza della biodiversità nei mercati finanziari. Nell'ecosistema dei mercati finanziari, l'esistenza di specie diverse di banche è un pregio, non un limite. In caso di crisi sistemica, è probabile che il parassita, il fattore di crisi, danneggi maggiormente alcune specie di banche piuttosto che altre. Qui invece si va nella direzione opposta, si punta alla standardizzazione: un mercato piatto, costituito in buona sostanza solo di banche SpA. Si è posto l'accento sulla contendibilità, come se fosse un valore in senso assoluto nel sistema creditizio. Io invece faccio mie le parole di un ex direttore centrale di Bankitalia, Angelo De Mattia: il fine di una banca non è la contendibilità, ma fare bene il credito e tutelare il risparmio. Si ritiene che alcune banche popolari non abbiano adempiuto con diligenza a tali compiti? Bene, colleghi, vi do una notizia: anche alcune banche SpA non l'hanno fatto, eppure non mi sembra che qualcuno abbia proposto di abolire tutte le banche SpA, anzitutto perché sarebbe un assurdo, ma soprattutto perché i colpevoli hanno sempre un nome e un cognome. Per sanzionarli esiste un'apposita autorità di vigilanza nazionale (tra l'altro, ne esisterà a breve anche una sovranazionale), che, anche in virtù dell'atto del Governo n. 147, attualmente in esame in Commissione finanze, godrà di tutte le facoltà necessarie per intervenire in caso di comportamenti scorretti. Se poi si va oltre, c'è la magistratura. Se invece il problema è la competitività delle banche popolari rispetto ad altri modelli bancari, allora che sia il mercato a decidere chi deve sopravvivere e chi deve sparire o cambiare e non già un atto forzato e illiberale. In un mercato competitivo che - certo - non sia viziato da irregolarità o accordi sottobanco, la concorrenza e la diversificazione dell'offerta sono un valore aggiunto che può portare solo benefici alla clientela. Potrei andare ancora avanti nello sfatare i tanti miti che hanno accompagnato questo decreto-legge. Potrei parlare dell'incredibile limitazione al diritto di recesso dei soci «anche in deroga alle norme di legge»

sede. In conclusione, ritengo che questo provvedimento avrà effetti esattamente inversi a quelli sperati: ulteriore allontanamento del sistema creditizio dall'economia reale, minore offerta al pubblico, minore diversificazione dei prodotti, minore resilienza sistemica e minore capacità di assorbire eventuali futuri *shock* finanziari. Se l'idea era quella di avvicinare domanda ed offerta creditizia e rendere la vita più semplice a cittadini e imprese, mi spiace, ma credo che i vostri conti siano totalmente errati e che, per dimostrare che questo Governo ha i numeri per fare ciò che vuole,

questo provvedimento si compone di 12 articoli. Su 11 articoli c'è un consenso piuttosto ampio e non stiamo parlando di cose di poco conto, perché parliamo del potenziamento del Fondo centrale di garanzia, del finanziamento alla piccola e media impresa, delle *start up* per le piccole e medie imprese innovative, dei finanziamenti al servizio delle esportazioni, del sostegno agli investimenti esteri che vengono in Italia; parliamo, nuovamente, di patrimonializzazione e di ristrutturazione delle imprese e anche di benefici fiscali sui marchi e sui beni immobiliari. C'è poi l'articolo sulle banche popolari. Credo che qui bisogna riconoscere il buon lavoro, che è stato svolto alla Camera dei deputati, di miglioramento e di integrazione del testo uscito a fine gennaio dal Consiglio dei ministri. né i deputati, né il Governo possiedono fino ad oggi la condizione costituzionale di approvare da soli e definitivamente una legge. Fintantoché esiste il bicameralismo, questo va rispettato e - aggiungo - non solo nella forma, che qui di fatto è rispettata, ma nella sostanza. Il Senato non è stato messo nelle condizioni di apportare modifiche ed integrazioni al provvedimento pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Questa condizione non è stata garantita né dal Governo, né dalla Presidenza di quest'Aula. Il mangiare questa minestra o saltare dalla finestra, dal momento che c'è il voto di fiducia, non depone a favore della serietà e della dignità delle istituzioni. Il Gruppo Area Popolare sostiene lealmente il Governo. Lo sostiene perché noi non vogliamo ricadere nella situazione di fine 2011; lo sostiene perché non dimentichiamo i segnali degli elettori nel 2013 e perché crediamo che la politica di riforme ed il sostegno al nostro apparato produttivo siano determinanti per la ripresa. Lo sosteniamo con responsabilità, anche in passaggi delicati, come è avvenuto la settimana scorsa, con le dimissioni del ministro Lupi. Questo non significa però celare le nostre critiche, rinunciare alle nostre proposte e alle nostre convinzioni. allora con franchezza che sulle popolari il Governo è stato quantomeno troppo zelante e troppo frettoloso. Il Governo Renzi aveva ed ha l'autorevolezza, la convinzione e le motivazioni per guidare alla luce del sole dei processi riformatori, per confrontarsi con le parti sociali e, possibilmente, per condividere le sue scelte con la maggioranza e, in questo caso, per rispettare l'articolo 41 della Costituzione e rafforzare al tempo stesso il sistema bancario italiano.

come tuteliamo gli impieghi verso le famiglie e le imprese italiane. È stato autorevolmente detto dal Governo che questa riforma avrebbe ridotto il numero dei banchieri e aumentato il credito alle piccole e medie imprese. Non ho questa certezza, quantomeno sul credito alle piccole e medie imprese. So che assecondiamo una scelta

da cui la necessità di adottare efficaci forme di Governo e un'elevata capacità di finanziamento delle banche; da qui, ancora, le modifiche all'attuale disciplina delle popolari. Non critico, in linea di principio, questa scelta tecnocratica della banca senza rischi, ma vorrei che la politica, in Europa e in Italia, si prendesse il suo spazio, per tutelare la democrazia economica o - se volete - l'economia sociale di mercato, per garantire la presenza concorrenziale di diverse tipologie di intermediari e creare rapporti virtuosi tra grandi banche e banche del territorio. Vorremmo cioè capire dal Governo se c'è una visione strategica sulle banche italiane, se essa coincide con quella dei regolatori o se vogliamo garantire un equilibrio del sistema - se vogliamo cioè un'impresa bancaria che abbia come sua finalità, da un lato, la tutela del risparmio, ma anche gli impieghi sul territorio - e se per rendere più competitiva la nostra economia si porrà mano - e in che modo - ai 185 miliardi di euro di sofferenze lorde delle banche italiane, oltre ai 350 miliardi di euro di crediti deteriorati, che pongono un limite al credito e alle famiglie. Ma dato a Cesare quello che è di Cesare, adesso parliamo delle popolari. Ho sentito in questa Assemblea, da colleghi preparati e che stimo, richiamare, per le popolari, l'articolo 45 della Costituzione Costituzione e la tutela costituzionale alle cooperative. Dico subito che per me le banche popolari sono un equivoco giuridico:

occorre la natura non speculativa della società, l'indivisibilità e l'indisponibilità del patrimonio e la non remunerazione del capitale. Domando dunque a voi, senatori e senatrici: può mai essere cooperativa un'impresa quotata in Borsa? Allora, il voto a testa diventa sì un orpello allo sviluppo capitalistico di quella banca popolare il paravento per singoli o per gruppi di potere che esercitano un controllo prolungato e incontrollato. Quindi, per noi il Governo fa bene a sciogliere questo nodo, *tertium non datur*: o società per azioni o vera cooperativa. Poi, questa forma ibrida, questo centauro può oggettivamente essere uno svantaggio competitivo sul mercato dei capitali? Banca d'Italia ci dice che il CET1, cioè il patrimonio di migliore qualità, è stato raggiunto all'ultimo minuto grazie a faticose misure di capitalizzazione da parte delle popolari.

a carico del Monte dei Paschi, 500 milioni della Carige, ma 3,7 miliardi sono probabilmente le perdite delle popolari italiane nel 2014. 2014. Ancora, essere banca del territorio significa che depositi e impieghi siano concentrati in misura rilevante in quel determinato e circoscritto territorio (per esempio, nelle banche di credito cooperativo, almeno il 95 per cento di impieghi, e ovviamente di depositi), mentre le

Lei sa che sono buono, se non mi provoca. e che italiano rimarrà sempre, rappresentato dalle banche di credito cooperativo. Dovremo preservare i valori della cooperazione, la prossimità al territorio delle banche di credito cooperativo; allora sì che ci dovremo impegnare per realizzare questo legame virtuoso tra risparmi risparmi del territorio e impieghi sul territorio. Infine, la difesa dell'italianità. Il rischio di scalate e di OPA ostili e totalitarie c'è, è inutile negarlo; però mi limito qui, adesso, in ad un'osservazione finale: se il nostro Paese vuole difendere e migliorare il proprio benessere, deve poter contare su un capitalismo nostrano più moderno, più pronto all'impegno negli investimenti nelle imprese e negli intermediari bancari piuttosto che nell'immobiliare - ieri in Italia, oggi all'estero - o nelle rendite finanziarie. Perché delle due l'una: o alziamo le barricate, blocchiamo le scalate, estere o italiane, e diminuiamo la capacità di capitalizzazione degli intermediari bancari - ma di tutte le nostre imprese - o apriamo ed eleviamo la capacità di finanziamento con rischi che ovviamente possono anche diventare opportunità (noi speriamo con l'accompagnamento del Governo). Noi scegliamo allora questa seconda opzione. Votiamo il decreto di 12 articoli;

ci troviamo oggi, 24 marzo, a discutere dell'ennesimo decreto-legge incostituzionale del Governo Renzi, scadente e in Il decreto, cosiddetto delle banche popolari, è stato assegnato alle Commissioni finanze e industria del Senato solo martedì 17 marzo. Abbiamo avuto pertanto tre giorni lavorativi per discutere un decreto che: modifica radicalmente l'impianto delle banche popolari; stabilisce tempi certi per la portabilità gratuita dei conti correnti; autorizza la Cassa depositi e prestiti all'esercizio diretto del credito; introduce la categoria delle PMI innovative; modifica la *patent box*; modifica la tassazione degli investitori istituzionali esteri inseriti nella *white list*; aumenta lo stanziamento delle garanzie statali per le imprese in amministrazione straordinaria; modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese; sopprime la possibilità da parte del CIPE di emanare delibere emanare delibere per interventi sul fondo di garanzia; stabilisce una corsia preferenziale per l'accesso al credito per le imprese che forniscono l'ILVA di Taranto. Mi sembrano pochini tre giorni per analizzare attentamente tutte queste cose. Ma forse la necessità ed urgenza del Governo Renzi era quella di porre la questione di fiducia e costringere la propria maggioranza a votare favorevolmente per questo decreto con la solita minaccia di elezioni anticipate. Non solo: in Commissione finanze, all'audizione dell'Associazione nazionale tra le banche popolari, abbiamo assistito - come oggi - all'intervento del senatore Luigi Marino, che non sapeva non sapeva se il suo partito sarebbe riuscito a modificare questo provvedimento ma ci avrebbe provato. Non abbiamo visto nessun emendamento a sua firma e oggi vota la fiducia. E che dire del senatore Azzollini, che si innervosisce perché alcuni emendamenti di Forza Italia sono stati ritirati e trasformati in un unico ordine del giorno, che non raggiunge però lo scopo di trovare una via di una via di fuga per la Banca popolare di Bari? Un insieme di atteggiamenti, più o meno leciti, per accattivarsi la *lobby* di turno, trasformando ogni decreto-legge o disegno di legge in un *puzzle* raffigurante Arlecchino, che sta tanto bene con Pinocchio. Come si fa a lavorare così? E lei, caro Renzi, non aiuta certo questo Parlamento con l'emanazione di continui decreti-legge al limite della costituzionalità.

faccia l'analisi dei decreti attuativi che devono essere ancora emanati e faccia lavorare i suoi Ministri. È inutile vantarsi di fare leggi se poi non possono essere attuate; come ha ricordato il suo ministro Boschi in quest'Aula, citando Fanfani, «in politica le bugie non servono». Ma torniamo a questo bel regalino postnatalizio. Sono note a tutti le indagini aperte dalla procura di Roma e dalla CONSOB per movimenti anomali dei titoli delle banche popolari, in special modo della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio; per non parlare del giallo sulla presenza della ministra Boschi a quel Consiglio dei ministri, collegata, per legami familiari e azionari, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, configurando un possibile conflitto d'interessi. Sarebbe utile, per dirimere ogni dubbio e riportare un minimo di trasparenza in questo Governo, visto e considerato ciò che è accaduto anche negli ultimi giorni, che il presidente Renzi, che sin dall'inizio del suo mandato ha più volte utilizzato la parola «trasparenza» nei suoi *spot* mediatici, senza mai attuarla, pubblicasse almeno il verbale del Consiglio dei ministri in questione. Avete giustificato, la necessità ed urgenza di questo decreto affermando che le banche popolari da anni dovevano essere riformate. D'altronde, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato segnalava questa necessità a luglio 2014, come pure la Banca d'Italia ad aprile. Suggerivano delle modifiche regolamentari, nessuna imposizione; il tutto per favorire la piena contendibilità degli assetti proprietari e il ricambio della compagine sociale. Da notare che nella nota del Servizio studi non si fa riferimento alla necessita di trasformazione in SpA Affermate, inoltre, che le banche popolari devono essere più competitive e appetibili, reperire capitali e concedere maggiori crediti alla clientela e rimettere, così, in moto l'economia nazionale. però, vi è sfuggita l'analisi degli ultimi tre anni. Infatti le banche popolari negli ultimi tre anni hanno realizzato aumenti di capitale per oltre nove miliardi di euro, senza bisogno di alcun decreto-legge. Hanno visto aumentare la loro provvista di oltre il 18 per cento, pari a 60 miliardi di euro, con un incremento del numero assoluto dei clienti del 6 per cento, pari a 700.000 unità. Come rilevato dall'Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, nel triennio 2010-2013, ossia in piena crisi economica, le banche popolari hanno aumentato di oltre il 15 per cento il credito concesso ai loro clienti, mentre le altre banche, nello stesso periodo, hanno diminuito hanno diminuito l'ammontare dei loro prestiti del 5 per cento circa. Alcune banche popolari hanno perso il loro spirito iniziale? È cambiata la loro natura cooperativa e di vicinanza al territorio? Regolamentiamole meglio, ma non facciamo di tutta l'erba un fascio. Secondo voi, bastano tre giorni, per valutare e analizzare tutte le conseguenze che queste modifiche al testo unico bancario avranno sulle nostre banche popolari? Forse non si è voluto accertare il vero impatto di queste modifiche, perché il vero intento del decreto-legge in esame è mettere alcune nostre banche popolari in mano agli speculatori finanziari, o forse salvarne altre. Infatti l'obbligo di trasformazione in SpA colpirà solo le banche popolari con un attivo maggiore agli otto miliardi, senza nessuna spiegazione. Infatti nella direttiva CRD IV (relativa alla vigilanza bancaria europea) si classificano le banche con attivi tra i 3,5 e 30 miliardi come banche intermedie e quelle con attivi inferiori ai 3,5 come banche minori. Ci sarebbero tante altre cose da dire solo all'articolo 1 del decreto e il tempo a mia disposizione sta per terminare. Concludo quindi con gli ultimi due articoli, l'8-*bis* e l'8-*ter*, altre due perle di saggezza di questo Governo. Con l'8-*bis* si elimina la possibilità da parte del CIPE di deliberare specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso, da parte delle PMI del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia. Con l'8-*ter* invece si riconosce la priorità di istruttoria e delibera per l'accesso al Fondo di garanzia, per le richieste effettuate da quelle imprese che forniscono beni e servizi all'ILVA di Taranto. Ossia, da una parte si taglia una via preferenziale per l'intero Mezzogiorno, dall'altra la si istituisce solo per l'ILVA di Taranto. Vorrei anche ricordare che la che la Toscana non può accedere al Fondo nazionale di garanzia per le PMI, ma questo non importa al *mister* Renzi. Questo Governo dimostra ancora una volta di avere due pesi e due misure, una visione dell'Italia al limite della schizofrenia

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 trasforma coattivamente in società per azioni le banche popolari con attivi superiori otto miliardi ed obbliga quelle con attivi inferiori a questa soglia a non superarla, pena la trasformazione forzosa in SpA. Perfino nelle banche popolari con attivo sotto sotto la soglia degli otto miliardi, e che dunque resterebbero cooperative, il passaggio al modello unico delle società per azioni è assai agevolato, sottraendo ai soci la determinazione delle maggioranze richieste e riducendo drasticamente i *quorum* assembleari per il passaggio dalla forma cooperativa alla SpA, anche fuori dai casi di esigenze di rafforzamento patrimoniale. Non si comprende, in primo luogo, come ampiamente emerso dai lavori parlamentari, quale sia la necessità e l'urgenza di intervenire con un decreto-legge sulle banche popolari, avendo peraltro tutte superato brillantemente gli esami della Banca centrale europea. Altrettanto incomprensibile è come si sia arrivati ad individuare la soglia di otto miliardi, che non trova riscontro in alcuna normativa esistente, primaria o secondaria, nazionale o internazionale. La nostra Costituzione non prevede certo limiti alla cooperazione, anzi, oserei dire che la incentiva quando fa comodo ad alcuni: quantomeno, se proprio si voleva indicare una soglia dimensionale, l'unica con un qualche crisma di oggettività è quella prevista dalla normativa europea per le banche vigilate dalla BCE, pari a 30 miliardi. Tale limite avrebbe pure l'ulteriore pregio, a differenza di quello prescelto, di consentire alle banche popolari rimanenti operazioni di ulteriore consolidamento e, soprattutto, di proseguire nell'erogazione di credito senza dover abbandonare la forma cooperativa. A questo proposito, mi sembra poi paradossale che si vada a riformare - ma sarebbe più appropriato dire cancellare - proprio il settore delle banche popolari che storicamente, ma specialmente negli ultimi anni di una crisi accresciuta dalle grandi banche - non dalle piccole - hanno di più aiutato e sono più state vicine alle piccole e medie imprese e alle famiglie. Pochi ed eloquenti dati: nel 2014 le banche del credito popolare, che occupano circa 82.000 persone, hanno erogato impieghi alle piccole e medie imprese per oltre il flusso dei nuovi finanziamenti alle piccole e medie imprese è aumentato di circa 30 miliardi di euro; alle imprese esportatrici sono stati erogati 42 miliardi di euro. La quota di mercato delle banche popolari nei sistemi economici a prevalenza di piccole e medie imprese è del il 33 per cento del resto del sistema. Ogni anno la categoria devolve a sostegno dei territori di riferimento circa 140 milioni di euro; nell'arco della crisi le donazioni

conoscenza e vicinanza dei territori - rischierà di produrre l'effetto contrario e cioè una stretta creditizia proprio nei confronti delle piccole e medie imprese, avvantaggiando solo gli speculatori e con pesantissime ricadute negative, anche da un punto di vista occupazionale. Una volta eliminata la struttura cooperativa delle banche popolari, infatti, queste saranno prevedibilmente facile preda degli speculatori, che non si preoccuperanno certo, né di finanziare le famiglie e le piccole e medie imprese - più rischiose - né di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

per l'occupazione, non dovrebbe avvenire attraverso questo decreto, ma da una riflessione condivisa, al fine di tutelarne il valore dimostrato, specie in questi anni difficili. Le situazioni incresciose hanno riguardato il sistema bancario italiano, europeo ed internazionale ed hanno coinvolto società di *rating* di fama internazionale, nonché una lunghissima lista di istituti finanziari globali: Lehman Brothers, Deutsche Bank, RBS, Socièté Generale, JP Morgan, Citigroup. Questi sono stati i fattori di crisi e di distruzione del risparmio, non certo le banche popolari del territorio. le banche internazionali sono state protagoniste dei misfatti dell'ultimo decennio, entrando nel capitale delle banche popolari acquisendone il controllo. L'evidenza scientifica ed empirica dimostra che le istituzioni finanziarie internazionali intervengono solo per fini speculativi. Per converso, le banche popolari, non solo non hanno mai creato problemi, ma sono state chiamate a risolverli. Lo strumento del decreto-legge, che vorrebbe essere varato con i requisiti di necessità e urgenza, in questo caso ha rappresentato un vero atto di arbitrio. Lo hanno confermato i pareri di autorevoli costituzionalisti, fra tutti costituzionale Cesare Mirabelli, già più volte citato, ma non è il solo. C'è un contrasto con l'articolo 77 della nostra legge fondamentale, ma ci sono, come ha rilevato intervenendo sulla pregiudiziale di costituzionalità la vice presidente del nostro Gruppo, senatrice Bernini, anche violazioni agli articoli 47 agli articoli 47 e 70 della Costituzione. Si attenta alla raccolta del risparmio, si interviene in maniera disomogenea su questioni diverse, per non trascurare poi i sospetti di speculazione che ci sono a carico di chi, avendo potuto conoscere prima di altri i contenuti del decreto, potrebbe aver agito con spregiudicatezza sui mercati finanziari. Si sono attivati a tal fine la procura di Milano e quella di Roma; sta svolgendo accertamenti la CONSOB; sono stati chiamati in causa finanzieri molto vicini alla Presidenza del Consiglio, come tutti sappiamo. Per non dimenticare le vicende, già ricordate in questo dibattito, della Banca dell'Etruria, ai cui vertici ci sono state persone molto legate ad esponenti di punta del Governo Renzi, che vengono, chiedono la fiducia e non hanno nemmeno l'umiltà di aspettare di ottenerla. Potrebbero almeno farci questa grazia. Dopo le vicende del Monte dei Paschi di Siena è ancora la Toscana l'epicentro di vicende bancarie inquietanti. Qualcuno si potrebbe essere arricchito. Dovremo attendere anni e anni per conoscere la verità, come sta avvenendo grazie ad alcune inchieste giudiziarie per le vicende speculative sui mercati finanziari del 2011, che ebbero riflessi anche sulle vicende politiche e democratiche di questo Paese, sulle quali chiediamo

Dovremmo parlare molto di più della Banca dell'Etruria e di tante altre cose di chi oggi al Governo dovrebbe spiegare e giustificare. Con questo provvedimento si parla di modernizzazione. In realtà, si mortifica l'economia dei territori. Un sistema creditizio che è stato più attento alle esigenze di artigiani, famiglie, piccole e medie imprese viene penalizzato. Si favorisce la colonizzazione del nostro sistema creditizio. Del resto, siamo un Paese in vendita. I cinesi si prendono la Pirelli, le banche internazionali hanno conquistato i nostri principali istituti di credito ed altri ancora sono pronti a ghermire le banche popolari. Una riforma di sistema andava fatta, ma bisognava discuterla in maniera serena e approfondita attraverso disegni di legge. Si violano parametri europei, si agisce con il consueto metodo del decreto-legge e della fiducia, impedendo un'analisi approfondita e seria di vicende complesse che, nell'interesse nazionale, dovrebbero essere esaminate

per converso, il modello di un'economia pianificata. In conclusione, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, come ha osservato anche Cesare Mirabelli, il limite di 8 miliardi è arbitrario e non trova alcuna condivisione in regole europee. Come ha sostenuto il professor Ainis, il decreto-legge, nella parte di riforma delle banche popolari, è viziato da irragionevolezza e irrazionalità. E anche Flick, un esponente di Governo con maggioranze di sinistra, nella sua versione di giurista ne ha stroncato i contenuti e la modalità. che voteremo contro la fiducia, voteremo contro l'ennesimo strappo alla Costituzione, voteremo contro un Presidente del Consiglio più dell'Etruria che della Toscana, voteremo per la libertà del credito, dell'impresa e dell'economia. *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, mi limiterò solo ad alcune considerazioni tenendo conto di quanto ascoltato nel dibattito in Aula. alla prima, è evidente che la discussione si sia concentrata soprattutto sul primo articolo, quello riguardante le banche popolari. Voglio, però, dare il giusto risalto alle altre misure contenute in questo testo, che sono altrettanto importanti. Si tratta di sostegno reale alle piccole e medie imprese, all'*export*, all'internazionalizzazione, alle *start up* e alla portabilità dei conti correnti. Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, Nuova Sabatini, *patent box* e fondi di credito sono solo alcuni esempi della volontà di tratteggiare una prima fase di politica industriale svincolata dalla logica dell'emergenza e dalla contingenza delle singole crisi di settore o di azienda, per rilanciare la competitività e, quindi, l'occupazione Per venire all'articolo 1, le ragioni per le quali si giustifica l'intervento del Governo sono sostanzialmente due. La prima: vi è una dimensione oltre la quale una banca che agisce nel mercato è diversa da una che ha una vocazione di tipo territoriale? Si possono dare molte risposte a questa domanda, ma quella che mi sembra più appropriata è che, sopra una certa dimensione, la natura stessa della banca, anche se in origine popolare, si trasforma *de facto* in una banca pienamente di mercato, destinata a competizioni più ampie, a processi di capitalizzazione più sofisticati e, quindi, ad una gestione del credito molto più ampia e diffusa. La seconda ragione è che i ritardi dell'autoriforma di questo sistema, più volte evidenziati da tutti in questi anni, a lungo andare hanno reso necessario un intervento come quello intrapreso dal Governo. In quest'ottica - come ha detto il sottosegretario Baretta l'impulso di autoriforma delle banche di credito cooperativo, che è la conferma che non vi è alcun atteggiamento contrario alla democrazia economica né alla partecipazione. Questi due elementi, ossia il valutare se sopra una certa dimensione vi è un cambio di natura, da un lato, e la relazione più rapida possibile ai ritardi accumulati, dall'altro, sono gli assi portanti del provvedimento. Possono essere opinabili, ma non sono incostituzionali. È legittimo che vi siano opinioni diverse, ma fino ad ora la discussione si è incentrata in gran parte sulla soglia degli 8 miliardi, proponendone altri in alternativa, ma mai omettendo l'esistenza di un problema da risolvere. Tale soglia è fissata su base consolidata per i gruppi bancari ed è calcolata rispetto al totale dell'attivo. Il primo criterio è coerente con il principio di neutralità della disciplina bancaria rispetto all'articolazione individuale o di gruppo dell'impresa. Il secondo, in riferimento al totale dell'attivo, è coerente con i più recenti sviluppi della regolamentazione finanziaria, che vide questa variabile insieme ad altre come un indicatore in grado di ricomprendere la complessità dell'intermediario e la sua rilevanza per la stabilità del sistema finanziario. La soglia numerica ha il pregio di essere chiara ed oggettiva, a beneficio della certezza del diritto. Il valore di 8 miliardi, inoltre, appare ragionevole alla luce dei dati, aggiornati alla metà dello scorso anno sulla dimensione delle banche popolari. Si può notare, infatti, come vi sia un salto netto fra le prime dieci con attivi almeno a doppia cifra - cercando, anche qui, di dare dati reali, e non quelli sbagliati che ho sentito nella discussione generale in riferimento a 160 miliardi - e le restanti 27 banche popolari. Il gruppo delle dieci maggiori comprende le sette popolari soggette alla vigilanza diretta del sistema unico europeo e tutte le quotate. La soglia di legge coglie, quindi, opportunamente la distinzione tra le due classi dimensionali. Inoltre, nel corso dell'*iter* alla Camera, com'è stato sottolineato, sono state apportate modifiche migliorative, come l'approvazione degli statuti, la soglia di diritto al 5 per cento, con una maggioranza inferiore di quella prevista dal codice civile, ed i La *ratio* del provvedimento, quindi, risiede nello stimolo ad agire rapidamente, e non solo per favorire un miglior controllo, ma anche per sviluppare gli elementi che mancano al nostro sistema per dirsi maturo. a nostro avviso il Governo ha messo in opera un passo in avanti nel miglioramento del sistema finanziario italiano, nessuna finanziarizzazione e nessun attacco alla democrazia economica. La riforma, oltre a facilitare il ricorso al mercato dei capitali da parte delle banche popolari, potrà anche migliorarne la gestione nell'interesse di tutta l'economia nazionale. Temere lesioni allo spirito cooperativo ed al legame stretto con un territorio, nel caso di grandi banche complesse, non solo è anacronistico, ma è in contrasto con la realtà dei fatti ed è inutile appunto forzare i dati a proprio piacimento. Conseguenze negative per l'occupazione, inoltre, discenderebbero dal mantenere gli istituti in una condizione di fragilità patrimoniale e gestionale, e non certo da un assetto societario che può, anzi, facilitare la ricerca di efficienza e di economie di scala. Altro che 20.000 posti di lavoro a rischio!

la spiegazione delle ragioni - ma perché lo suggerisce il buonsenso. La nostra economia, le nostre imprese hanno bisogno di banche efficienti, patrimonialmente solide, a loro agio nel mercato internazionale; banche che siano in grado di accompagnare, anzi di sollecitare la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione delle imprese più dinamiche, crescita da cui dipende molta parte del nostro futuro; banche che vivano nella concorrenza e siano in grado di favorirla. In questo senso, mentre capisco l'imbarazzo di chi spesso ha usato le banche per altri fini, mi stupisce il comportamento di alcune altre forze politiche, il voler confondere la riforma della *governance* con il ruolo verso le imprese e le famiglie. Avremo ancora bisogno di banche piccole e cooperative, che sappiano però interpretare i migliori valori di comunità che i territori sanno esprimere, non dannosi e finti localismi, al servizio del tessuto dei risparmiatori e delle imprese che restano piccole; ma anche loro dovranno adoperarsi per trovare soluzioni organizzative che le rendano più sane ed efficienti. Il dibattito ha visto una contrapposizione spesso aspra, su posizioni legittime ma differenti. Voglio solo rivolgere un richiamo personale, a me stesso e a tutti i colleghi, in particolare al senatore Crosio: c'è uno stile che dovrebbe riguardare tutto il Parlamento, maggioranza e minoranza, oltre il confronto, la dialettica politica e il merito delle questioni.

la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1813, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

accolto, limitatamente a comprovate esigenze di natura fisica ed istituzionale, alcune richieste di votare per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

votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1813, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

il sogno di un ragazzo, che stava per andare a giocare una partita con i suoi amici, si è spezzato a causa di un incidente provocato probabilmente da un pirata della strada dopo il disastro combinato, è scappato; anche se le ultime notizie di stampa dicono che si è costituito, pur ammettendo parziale verità. Sarà poi chi è competente ad indicare le responsabilità dei fatti.

benché abbia commesso omicidi così efferati - voglio già iniziare a chiamarli così - il giorno dopo può circolare liberamente con la sua patente e riproporre probabilmente gli stessi pericoli a chi, invece, accompagna il figlio, in una giornata felice, ad una partita di pallone, ad un momento di spensieratezza. Occorre una riflessione di tutta l'Aula. Siamo probabilmente alle soglie dell'arrivo in Aula di questo provvedimento